una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, il Presidente della Repubblica, con decreto in data 30 agosto 2013, ha nominato senatori a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, il maestro Claudio Abbado, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo artistico e sociale, la professoressa Elena Cattaneo, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale, l'architetto Renzo Piano, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo artistico e sociale, il professor Carlo Rubbia, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale. A nome mio personale e dell'Assemblea del Senato, rivolgo il più cordiale e caloroso benvenuto ai nostri

Il senatore Claudio Abbado ha fatto sapere che, suo malgrado, non potrà prendere parte alla seduta odierna a causa di un'indisposizione. Con l'augurio di una pronta guarigione, rivolgo anche a lui le congratulazioni per la nomina a componente di questa Assemblea.

L'ordine del giorno G1 è accoglibile nella sua interezza, nel senso che il Governo non solo è ben conscio dell'importanza di affrontare questa tematica con spirito programmatorio, anche al fatto che si sia trovato un intento unificatorio nel proporre stimoli al Governo per agire nel senso di una corretta programmazione di reperimento delle risorse e di tutto quanto possa portare ad affrontare in maniera costruttiva questo grande problema.

le mozioni che oggi abbiamo affrontato - su questo insisto molto - hanno un'importanza notevole, perché

in modo molto chiaro e preciso, di una svolta radicale nel campo della difesa del suolo. Non è più tempo di

che il nostro sistema territoriale, i nostri fiumi, il nostro paesaggio e il nostro suolo sono un bene comune e - vorrei ricordarlo ancora una volta - un bene tutelato tutelato anche dal punto di vista costituzionale. Su questo quindi bisogna essere coerenti oggi, nel momento in cui ci si assume una serie di impegni. Come

È necessario intervenire per cambiare completamente quella che è stata la strategia fino ad oggi, una non strategia che ha fatto sì che per ogni miliardo investito nella prevenzione ne sono stati spesi 100 per riparare a tutti i danni, i danni, intervenendo in emergenza. Proprio il cambio di strategia e il considerare la messa in sicurezza e la difesa del suolo come l'opera prioritaria del Paese significa anche fare una scelta economica chiara e precisa che frutterà, e potrà fruttare molto di più in termini occupazionali. Lo ricordava qualcuno nel dibattito di questa mattina: se andiamo a confrontare il numero di posti di lavoro sviluppati per una grande opera infrastrutturale e quelli che potrebbero nascere - sono numeri che abbiamo già a nostra disposizione - dalle piccole e medie opere di intervento per la messa in sicurezza, non c'è paragone.

chiudere una volta per tutte con i tentativi, che pure sono stati fatti anche recentemente, di portare avanti altre sanatorie. L'abusivismo è stato un flagello per questo nostro Paese. È necessario farla finita una volta per tutte con le deroghe urbanistiche, che hanno permesso, pur con l'approvazione di piani di assetto idrogeologico, di continuare a rilasciare permessi per costruire in aree pericolose. I dati li abbiamo visti questa mattina: vi è quasi il 10 per cento del territorio nazionale che è a rischio. Vorrei qui ricordare al Sottosegretario per l'ambiente che questa questione non possiamo affrontarla soltanto nella dimensione del dissesto e della difesa del suolo. Dobbiamo sapere con chiarezza che gli eventi estremi aumenteranno nel nostro Paese, perché i dati sui cambiamenti climatici sono importanti e pesanti, e quindi bisognerà mettere in campo non soltanto il piano pluriennale, non solo il fondo per la per la difesa del suolo e quindi allocare risorse adeguate, ma bisognerà ricordarsi che è necessario avere una politica coerente di contrasto ai cambiamenti climatici. È una questione che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, lo vorrei ricordare proprio qui, in quest'Aula, perché nella scorsa legislatura al Senato - ahimè - fu approvata addirittura una mozione che negava i cambiamenti climatici. Credo che i dati siano oggi sotto gli occhi di tutti. Sono sempre più allarmanti e il nostro territorio, come sappiamo, è già particolarmente fragile per i tutti i motivi Quella delle risorse è una questione molto importante: avevamo chiesto un piano pluriennale; speriamo che almeno il fondo istituito possa essere rinforzato e che possano essere allocate le risorse adeguate.

per cui il giorno dopo delle disgrazie se ne discute e dopo 48 ore tutti i decisori politici dimenticano completamente. Spero che il dibattito di oggi possa segnare davvero una svolta da questo punto di vista.

sia nella precedente legislatura che in questa sono stati svolti dibattiti ed approfondimenti che hanno messo in evidenza una realtà disastrosa del Paese in ordine ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Una vera emergenza nazionale, certamente legata alla particolare conformazione del territorio, ma soprattutto all'antropizzazione dello stesso, all'abbandono dei terreni montani, all'edificazione spesso abusiva e talvolta anche irresponsabilmente autorizzata nelle aree a rischio di frana, di smottamento e di esondazione. Un'emergenza collegata anche al disboscamento, alla mancata pulizia dei boschi, della manutenzione dei versanti e dei corsi d'acqua. Le conseguenze dell'esposizione al rischio sono state e continuano ad essere drammatiche, sia in termini di perdita di vite umane, sia in termini di danni ambientali ed economici, che richiedono risorse ingenti per poterli affrontare. Nella scorsa legislatura sono stati fatti passi importanti per definire, in accordo con le Regioni, un piano per contrastare i dissesti idrogeologici, purtroppo però senza risultati concreti, nonostante lo stanziamento di quasi 2,5 miliardi di euro da parte dello Stato e delle Regioni. Da parte del precedente Governo sono state anche tentate delle linee strategiche per il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, per la gestione sostenibile e per la messa in sicurezza del territorio, ma di fatto queste non sono state ancora messe in pratica. Il piano di emergenza essenziale riguarda la costituzione di un'autorità di bacino distrettuale ed il divieto dell'uso ai fini residenziali e produttivi o per servizi e infrastrutture delle zone classificate R4 (area a rischio idrologico molto elevato),

sono stati valutati 40 miliardi per quindici anni, con circa 2,5 miliardi l'anno. Ma non basta: occorrono un salto di qualità e la consapevolezza che l'ambiente è un bene primario necessariamente da tutelare e per il quale bisogna investire. È comunque di tutta evidenza che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, oltre a perdere ulteriore credibilità rispetto ad altri Paesi (e magari anche aiuti dall'Unione europea per inadempienza rispetto al mancato recepimento delle direttive in materia), sarà sempre più difficile ed insostenibile far fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali. Secondo il Gruppo della Lega Nord, occorrono impegni precisi da parte del Governo per restituire un fondo nazionale atto a finanziare un programma organico in tema di difesa del suolo e di prevenzione dei dissesti idrogeologici, privilegiando dunque la logica della prevenzione rispetto a quella delle gestione dell'emergenza. Certamente occorrono interventi immediati per finanziare ed affrontare le situazioni a più elevato rischio idrogeologico a salvaguardia della sicurezza del patrimonio ambientale e culturale, ma anche delle infrastrutture che sono strategiche per lo sviluppo, evitando però sistemi centralizzati di gestione degli interventi e facendo ricorso al principio di sussidiarietà, capace di coinvolgere positivamente Comuni, Province e Regioni, nonché imprese agricole e forestali. Come ha sottolineato anche il ministro Orlando nell'esposizione delle sue linee programmatiche lo scorso 25 giugno, occorre sbloccare le risorse già previste nella precedente legislatura a seguito degli accordi di programma sottoscritti con le Regioni per interventi prioritari di prevenzione del dissesto. Occorre poi adottare tutte le iniziative possibili per escludere dai vincoli del Patto di «stupidità» interno le risorse che i Comuni e le Regioni destinano agli interventi dal Gruppo* *LN-Aut**).* Va inoltre ribadito e sottolineato che i veri conoscitori dello stato di salute del territorio e delle relative necessità di intervento per la messa in sicurezza e per la prevenzione dei rischi dei pericoli derivanti dalle calamità naturali sono gli amministratori locali. È dunque opportuno mettere gli stessi amministratori e i loro volontari al centro al centro delle attività relative all'individuazione, alla predisposizione e all'esecuzione degli interventi di mitigazione allo scopo censiti. Appare quindi necessaria una revisione delle norme vigenti in campo di prevenzione e di lotta al dissesto idrogeologico, eliminando le disposizioni che, di fatto, rendono farraginose le procedure atte all'esecuzione degli interventi ed all'assegnazione delle risorse medesime. Tutte le mozioni presentate dai Gruppi, pur caratterizzandosi per un proprio approccio e una propria sensibilità, concordano nell'analisi del problema, sulla necessità di intervenire rapidamente su alcuni punti fondamentali e strategici e su diverse proposte per affrontare i problemi in linea preventiva e con finanziamenti concreti. Inevitabile - e dunque positivo - è lo sforzo profuso per giungere

Le mozioni, su cui in mattinata è stata avviata un'intensa discussione, si collocano in un percorso parlamentare e normativo che - sebbene ampio - ancora non ha condotto a riscontri fattivi, come purtroppo l'attualità ci continua a confermare. La questione o, meglio, il problema della tutela del territorio e della lotta al dissesto idrogeologico riemergono in maniera ciclica all'attenzione del Paese, con l'inevitabile seguito emergenziale che questo comporta e che, di fatto, sembra voler legittimare una forma di elusione di qualsiasi piano di intervento programmatico e lungimirante. Sono volutamente critico. Questo purtroppo sembra voler confermare che la lotta al dissesto idrogeologico non sia una priorità per questo Paese, anche se le buone intenzioni, a seguito di eventi calamitosi, sembrano testimoniare tutt'altro. i vincoli di bilancio, infatti, si continua a non considerare prioritarie le politiche di manutenzione preventiva del territorio finalizzate ad impedire eventi calamitosi. Spesso dinanzi ad una tragedia, per così dire ambientale, quello che emerge è la mancanza di una responsabilità chiara, accompagnata da polemiche verso questo o quell'ente. E si ritorna sempre sulle colpe ataviche del Paese: assenza di investimenti infrastrutturali finalizzati alla manutenzione delle aree a rischio, a cui si aggiunge la mancata applicazione delle norme in materia di lotta all'abusivismo edilizio. Ciò si unisce ad una certa - permettetemi di dire - cialtronaggine amministrativa che rende il tutto ancora più complesso. Gli eventi calamitosi che si sono susseguiti negli ultimi anni in Italia hanno sottolineato al Paese intero che non esistono zone esenti da rischio, quasi a conferma del fatto che in Italia, ben prima di qualsiasi mancato intervento o di cattiva prassi, esiste una diffusa cultura dell'illecito. Il dramma di questi mesi sottolinea la debolezza del territorio italiano, unita alla palese debolezza gestionale e amministrativa del nostro Paese nel salvaguardare il territorio. Come viene più volte ripetuto nelle mozioni di tutti i Gruppi, il suolo è un bene irriproducibile ed essenziale che va tutelato, proprio perché legato ai processi ecologici che, se intaccati, possono compromettere gli equilibri della biodiversità e dell'ambiente. Infatti, dai cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo e dalla consapevolezza che gli impatti che essi determinano sono destinati a crescere in maniera esponenziale deriva la necessità di affrontare i problemi ambientali con strumenti nuovi e adeguati che si basano su altrettanto adeguate e certe risorse economiche. Ma in Italia, oltre ai problemi di carattere tecnico, esistono anche e soprattutto forti limiti amministrativi, legittimati da vistosi tagli di bilancio operati nei confronti del Ministero dell'ambiente, che negli ultimi quattro anni ammonterebbero a circa il 90 per cento delle disponibilità. Io stesso ho provveduto a denunciarlo in diversi atti parlamentari nella scorsa legislatura. Nel 2009 veniva annunciato il decollo del piano straordinario per combattere il dissesto idrogeologico e la promessa da parte dell'allora Governo di circa 2,5 miliardi per finanziarlo; si trattava di risorse orientate alla messa in sicurezza delle aree più a rischio. Non dimentichiamo che nella manovra di agosto 2011, però, è stato operato un taglio di 500 milioni di fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Nella legge di stabilità 2011 ammontavano a circa 6 miliardi di euro i tagli operati dall'allora Governo al Ministero dell'ambiente, con il rischio di vanificare ogni progetto o iniziativa orientata alla tutela dell'ambiente e svuotando di fatto l'utilità del medesimo Dicastero. Abbiamo assistito in Italia al consolidamento della filosofia del «taglia e cuci», dove ai tagli indiscriminati e irrazionali a cui conseguono tragedie annunciate ed evitabili, si accosta una gestione pressappochista dell'emergenza con l'erogazione rapida di risorse, le stesse che, erogate a tempo debito, unite a una maggiore lucidità da parte degli amministratori, avrebbero senz'altro impedito l'emergenza stessa. stessa. In una fase come questa il pressapochismo dovrebbe essere sostituito dalla razionalità funzionale degli enti locali. Avevamo sperato che con il piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio, presentato dal ministro Clini al CIPE lo scorso dicembre, sarebbe stato possibile fare un passo avanti. Ma al momento il piano resta in *stand-by*, a quanto pare per mancanza di risorse. Il piano definisce le linee guida e le misure per prevenire i rischi e i danni ai quali è sempre più esposto il Paese; risponde anche all'impegno del nostro Paese nell'ambito della direttiva europea sulle alluvioni. Il piano prevede 2,5 miliardi l'anno di investimenti, di cui 1 miliardo di risorse pubbliche e 1,5 miliardi di risorse private agevolate con credito di imposta. Sarebbe necessario che gli investimenti pubblici per l'attuazione del piano fossero liberati dal vincolo del Patto di stabilità, in attuazione del criterio - condiviso tra l'altro dalla Commissione europea - secondo cui l'adattamento ai cambiamenti climatici deve rappresentare una misura strutturale per la crescita. l'ordine del giorno presentato insieme al collega Dalla Zuanna al decreto-legge n. 43, cosiddetto decreto emergenze ambientali, ed accolto dal Governo nel maggio scorso, si colloca proprio in questa direzione. Il Governo si è impegnato infatti a valutare la possibilità di predisporre, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», misure volte a consentire la deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno per le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per pagamenti relativi ad investimenti in materia di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici. Questo Governo sta dimostrando pragmatismo, oltre che una valida continuità con quanto operato dal Governo Monti, deve dare seguito agli impegni già assunti e trasformarli in piani operativi realmente attuabili. Deve trasformare le politiche di lotta al dissesto idrogeologico da accessorie a prioritarie. Appare opportuno ricordare che il *premier* Letta, nel suo discorso di insediamento alle Camere, lo scorso 29 aprile, ha sottolineato che «abbiamo un impegno alla prevenzione con piani straordinari di manutenzione contro il dissesto idrogeologico e la lotta all'abusivismo», mettendo dunque l'accento su un rinnovato impegno verso tali questioni. Voglio ulteriormente evidenziare che, nel solco di quanto operato dal Governo Monti, è possibile recuperare iniziative ed attività valide, capaci proprio di rinnovare questo impegno del Governo. Infatti, vale la pena ricordare che lo scorso settembre 2012, l'allora ministro delle politiche agricole Catania aveva presentato un disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo, nato proprio dall'esigenza di arrestare il fenomeno della cementificazione nel nostro Paese. In questa prospettiva ricordiamo che il ministro Orlando nei giorni scorsi ha presentato un disegno di legge recante misure finalizzate a rendere più agevole la demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree caratterizzate da elevato rischio idrogeologico. Per il 2013 è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per quei Comuni che facciano richiesta di risorse finalizzate all'abbattimento di immobili abusivi, consentendo in tal modo una semplificazione delle dinamiche di progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio. In tale scenario le mozioni in esame rappresentano sicuramente un ulteriore passo in avanti per garantire che tali temi vengano inseriti in maniera urgente nell'agenda politica nazionale con un'assunzione generale e condivisa di responsabilità da parte di tutte le forze parlamentari. L'obiettivo è dunque quello di puntare a un programma integrato di risorse, che renda attuabile il piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio, rinnovandolo e adeguandolo alle fattispecie calamitose che sono andate delineandosi negli ultimi mesi. È fondamentale, in questa fase, destinare risorse per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del territorio, che non possono assolutamente prescindere dalla definizione di un piano organico di gestione, prevenzione e difesa del territorio nonché di monitoraggio e controllo locale delle diverse e articolate specificità territoriali. Pertanto, consapevole del carattere urgente e indifferibile di questo rinnovato impegno verso il Paese e avendo piena fiducia nell'operato del ministro Orlando e di tutto il Governo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Scelta Civica all'ordine del giorno unitario. *(Applausi

quindi coerenti con una visione complessiva (non finanziamenti a pioggia), perché tante piccole opere producono molto più lavoro. Realizzando tante piccole opere mettiamo quindi in funzione una economia diffusa, anche perché tante piccole opere fanno lavorare magari imprese locali,

Andando nello specifico, nella nostra mozione abbiamo provato a far qualcosa di diverso, abbiamo provato ad individuare dei punti specifici. Il tema del dissesto idrogeologico, anzi del dissesto idrico e geologico, è molto vasto ma noi dobbiamo iniziare ad avere il coraggio di dire al Governo dove intervenire,

Bello. Bastava scrivere - perché in italiano più chiaro - che non si fanno condoni e si abbatte ciò che è abusivo. L'italiano è una bella lingua perché ci permette di essere chiari e definiti, altrimenti continuiamo ad usare usare un linguaggio non chiaro. A noi piace il linguaggio chiaro perché siamo persone dirette e vogliamo che la gente capisca; invece, se scriviamo in questo modo, usiamo quello che quando eravamo fuori chiamavamo politichese. Non vorremmo ancora del politichese.

c'è stata un'era, la famosa era Bertolaso, in cui la protezione civile ha fatto ben altro rispetto a quello che doveva fare. Vi è poi la parte sull'assicurazione da rischi naturali. L'assicurazione è una cosa che tutti i cittadini possono fare: volendo, un cittadino o un condominio si assicura. Siccome ho sentito dire che non c'è la possibilità di assicurarsi, vorrei dire oramai quasi dieci anni fa, in Afghanistan con Emergency; sono stato a fare la mia azione di volontario, anzi di cooperante, ed ero assicurato contro i rischi di guerra: era il 2003, due anni dopo l'uccisione di Massoud. E se hanno assicurato me, un cooperante, per i rischi da guerra, credo che sia possibile assicurare una casa in una zona a rischio. valutiamo l'opportunità di assicurare, quindi diamo ai cittadini la facoltà di assicurarsi.

Per quanto riguarda la nostra mozione n. 138, noi accogliamo la riformulazione che ci ha chiesto il Governo.

di gestione forestale; mi rendo conto che ci sono impegni finanziari, però avremmo voluto qualcosa di più; tuttavia ci accontentiamo, perché nella nostra mozione ci sono punti specifici dove chiediamo di intervenire, ed è interessante pensare di aiutare il Governo. Noi vorremmo aiutare il Governo a capire dove intervenire. Questo è il nostro piccolo auspicio, che è grande perché in questo modo noi diamo un aiuto al Governo a fare quello che deve fare, cioè eseguire la volontà del Parlamento. È bello pensare che il Governo esegua la volontà di noi parlamentari, perché altrimenti il Governo che deve fare? Decide lui? E noi che facciamo, ratifichiamo le sue decisioni? E quand'è che ci riappropriamo della nostra capacità di scegliere? Vogliamo scegliere, vogliamo decidere una volta per tutte di scegliere? Scegliere, infatti, significa accontentare qualcuno e scontentare qualcun'altro, ma il compito della politica è avere il coraggio di scegliere. Quindi noi vi chiediamo di votare a favore della mozione n.

signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, con l'ordine del giorno di cui abbiamo discusso e che è stato illustrato anche nell'intervento del Sottosegretario si chiede al Governo di avviare una nuova politica di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro Paese.

oltre 5 milioni di cittadini italiani sono esposti al pericolo di frane e alluvioni; la superficie del territorio italiano ad alta criticità idrogeologica è pari a quasi 30.000 chilometri quadrati, ovvero un decimo della superficie del nostro Paese. Conseguentemente, il numero delle vittime delle attività umane colpite dal dissesto idrogeologico è in costante e preoccupante aumento. Sembra un esercizio inutile ripetere

per effetto di scelte sbagliate e di programmazioni lacunose, non certo riferibili agli ultimi anni, ma risalenti e stratificate nel tempo. Sulla base di tali considerazioni è compito del Governo, ma deve essere scrupolo anche del legislatore, ripensare la strategia complessiva sulla soluzione dei problemi connessi al rischio idrogeologico nel territorio italiano. In tal senso l'ordine del giorno stimola il Governo e gli chiede una serie di impegni con la finalità di compiere un *reset* rispetto alle politiche del passato. Tra gli obiettivi di tale iniziativa va sicuramente ricompresa la necessità di realizzare una nuova *governance* delle azioni a tutela del territorio. In tal senso è necessaria una riflessione sull'attuazione e l'applicazione dei piani di assetto idrogeologico nei diversi bacini istituiti nel nostro A tale riguardo non si potrà non osservare che la relazione tra autorità di bacino ed enti locali non si è ancora pienamente realizzata e che gli stessi strumenti di pianificazione sono spesso stati emanati ed applicati in un clima di conflittualità e magari con il vizio genetico di studi e analisi tecniche non sempre rispondenti alle reali situazioni del territorio o, comunque, nella migliore delle ipotesi, non aggiornati. Proprio per questo ci si propone di riaffermare l'esigenza di una regia unitaria, con ciò non intendendo la volontà di favorire un neocentralismo di stampo meramente burocratico, bensì l'intento di superare la frammentazione creata dal diverso livello di competenze cui contrapporre invece una piena ed efficiente attuazione delle politiche di tutela del suolo e delle acque, affidandole alle autorità di bacino e alle Regioni. Altra priorità presa in esame dal documento posto alla votazione odierna dell'Aula è quella di incrementare la spesa dello Stato e delle Regioni per azioni ed iniziative di prevenzione e tutela del rischio idrogeologico. È stato detto da chi mi ha preceduto che i fondi assegnati per tale obiettivo sono oggettivamente insufficienti e spesso sono stati spesi con colpevoli ritardi, anche in modo farraginoso. Pertanto sarà necessaria, già dalla legge di stabilità per il 2014, la previsione di risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione e manutenzione ordinaria del territorio, raccordando gli stessi con i piani di bacino e con le scelte adottate dalla Conferenza Stato-Regioni-enti locali. Sarà altresì necessaria - l'ordine del giorno affronta detta esigenza in modo profondo e appropriato l'istituzione di un fondo nazionale per la difesa del suolo e la riduzione del rischio idrogeologico con il quale concedere risorse certe - molti interventi si sono

Spesso è molto più subdola ed ingannevole una deroga urbanistica munita di tutti i pareri e le autorizzazioni che non un abusivismo edilizio più facilmente ravvisabile e oggetto magari di procedimenti penali ed amministrativi rispetto ai quali dobbiamo solo auspicare un'accelerazione nella conclusione e non misure aggiuntive. Un altro impegno che si chiede al Governo con il presente ordine del giorno è quello di prevedere interventi di carattere normativo ed amministrativo finalizzati ad una maggiore integrazione della pianificazione urbanistica con le opere di difesa del suolo, raccordando piani urbanistici comunali e piani di area vasta con le esigenze solo strettamente collegate alla difesa del suolo. Si chiede altresì di dare pronta attuazione al piano straordinario per la difesa del suolo, con il quale siano stanziati finanziamenti per 2,5 miliardi di euro comprendenti fondi statali e regionali. Nell'ordine del giorno si pone l'ulteriore obiettivo della valorizzazione naturalistica dei fiumi come nuovo approccio e nuovo metodo per gestire e, soprattutto, prevenire le alluvioni che negli ultimi decenni hanno assunto dimensioni sempre più notevoli. Si evidenzia, come è stato ribadito da più senatori, il ruolo e la funzione dei consorzi di bonifica, il cui *know-how* può rivelarsi decisivo per serie ed efficienti strategie di prevenzione. Nell'ordine del giorno si fa anche riferimento e si auspica la valorizzazione ed un migliore coordinamento della protezione civile in concomitanza con eventi tragici dovuti al fenomeno di cui stiamo parlando. Questi in estrema sintesi i tratti salienti del presente ordine del giorno. Si tratta per il Governo di un'agenda ben definita cui informare ed adeguare le attività dell'Esecutivo e del Parlamento per i prossimi anni. Si tratta inoltre di obiettivi che suscitano largo consenso e che, se ben realizzati, potranno far voltare pagina al nostro Paese che non sarà più il tetro scenario di periodiche e luttuose tragedie, ma offrirà un modello di efficienza e di capacità nella soluzione di problemi così complessi. Proprio per queste ragioni, convintamente, annuncio il voto favorevole del

vorrei sottolineare l'importanza e il significato che assume la discussione di questo argomento oggi, proprio nei giorni in cui il Governo è impegnato nella predisposizione della legge di stabilità, perché sono fermamente convinto che l'ambiente e la difesa del nostro inestimabile patrimonio paesaggistico debbano essere inseriti tra gli interventi prioritari per il rilancio del nostro Paese. Questa è una proposta, un pensiero lungo, che ancor prima di tradursi in azione politica, deve realizzarsi nella società come acquisizione di un nuovo modello culturale. Deve diffondersi sempre più la consapevolezza che la bellezza del nostro patrimonio ambientale, che ci contraddistingue a livello internazionale, è la forza più importante che abbiamo e, al tempo stesso, di quanto esso sia fragile e vittima del disinteresse dell'uomo. Come ricordava il senatore Vaccari, negli ultimi decenni l'assenza di un'adeguata pianificazione territoriale ha portato ad un progressivo aumento della cementificazione. Inoltre, il sempre più diffuso ricorso alla pratica dell'abusivismo, le continue deroghe alla normativa urbanistica e le ricorrenti politiche di condono edilizio hanno impedito la creazione di una cultura diffusa in materia di sicurezza del territorio, di rispetto delle regole e di salvaguardia del suolo. Vorrei che tutti noi iniziassimo a pensare alla tutela e alla manutenzione del nostro territorio come la prima opera pubblica del Paese, sulla quale investire. L'Italia ha bisogno di tornare a crescere e di creare occupazione, soprattutto per i giovani, e la *green economy* - in assoluto il settore con prospettive più serie e durature di crescita - deve diventare il volano dove destinare parte dei risparmi derivanti dal rientro dalla procedura d'infrazione comunitaria per *deficit* eccessivo. Intendiamoci: è fuorviante pensare di farlo senza il passaggio dall'approccio dell'intervento *una tantum* e della sola risposta all'emergenza a quello della pianificazione e della programmazione di politiche di prevenzione nella gestione del territorio. Un euro speso in prevenzione ne fa risparmiare quattro in interventi di emergenza successivi ad eventi calamitosi come frane, alluvioni, allagamenti. Senza parlare della possibilità concreta di salvare vite umane. Inoltre, la mancanza di una *governance* unitaria, con la conseguente frammentazione e sovrapposizione delle competenze tra diversi soggetti e strumenti operativi, non solo rende inefficiente il sistema di pianificazione, gestione e monitoraggio degli interventi, ma non consente di pervenire ad una facile identificazione delle responsabilità.

la definizione di un percorso che porti all'individuazione di enti che, oltre a programmare interventi, abbiano le risorse necessarie per l'attuazione degli stessi. Non si può parlare di eliminazione dei sovralluvionamenti, di dragaggi nei tratti focivi dei fiumi, di taglio selettivo della vegetazione, di arginature, casse di espansione, se non sappiamo chi, oltre che pianificarle, deve occuparsi della loro attuazione e con quali risorse a disposizione. Chiediamo, quindi, l'eliminazione dei conflitti tra competenze e la semplificazione delle procedure decisionali. Bisogna dare sicurezza e certezza del diritto ai cittadini che hanno subito danni o, peggio, hanno perso la casa o la propria attività. Per questo, trovo più che doverosa la richiesta di promuovere forme di assicurazione da rischi naturali per cittadini ed imprese che implichino il coinvolgimento obbligatorio dello Stato. È prioritario, inoltre, restituire forza, dignità e autonomia, soprattutto finanziaria, al Dipartimento della protezione civile. È paradossale che esso venga lasciato senza risorse per operare in modo tempestivo ed efficace nel campo del contrasto ai danni provocati dalle calamità naturali. Nello stesso tempo, è più che opportuno valorizzare anche il volontariato e le squadre di protezione civile comunali. Ho potuto apprezzarne personalmente la generosità e la competenza: raro esempio civico che deve essere coltivato e sostenuto. Come devono essere promosse, per la manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua, soluzioni creative che rechino forme di incentivazione della partecipazione attiva della popolazione, anche mediante la sperimentazione di progetti che coinvolgano i lavoratori temporaneamente beneficiari di ammortizzatori sociali e i detenuti. Per quanto riguarda il tema specifico della difesa del suolo e del rischio idrogeologico, sono convinto che non sia più procrastinabile il cambiamento del nostro modello di sviluppo, che deve necessariamente basarsi: sulla scelta strategica della destinazione d'uso del territorio; sulla ricostruzione ecologica dei corsi di acqua, con una particolare attenzione ai programmi di manutenzione degli alvei fluviali, sempre più mirati a ridurre il rischio di alluvioni e a migliorare lo stato ambientale; e sul monitoraggio delle situazioni a rischio. Dobbiamo contrastare il disboscamento e l'abbandono dei terreni e riconoscere il valore strategico dell'agricoltura: non solo come presidio e strumento di manutenzione ordinaria del territorio, valorizzando la funzione dei consorzi di bonifica, ma anche e soprattutto come strumento per favorire l'occupazione giovanile. *(Brusìo. Richiami del Presidente).* E qui, consentitemelo, colleghi senatori, è giusto chiarire un aspetto non secondario nelle decisioni che saremo tenuti a prendere. Molte volte, io dico giustamente, si evidenzia come causa del dissesto idrogeologico l'eccessiva cementificazione, mentre sottovalutiamo un aspetto che è altrettanto determinante: l'abbandono del territorio agricolo, soprattutto quello collinare. La nobile pratica agricola, con la cura dei versanti, del bosco, delle sistemazioni idrauliche care al contadino, riusciva a mantenere salda e sicura la nostra collina. Quando si chiede un intervento per la prevenzione, penso sia importante creare un sistema di agevolazioni finanziarie, fiscali per il recupero dei coltivi, per la ristrutturazione di quei paesi che hanno subito un esodo agricolo e per far rivivere complessivamente le comunità, che sono un elemento fondamentale di forte contrasto al depauperamento del nostro territorio. la capacità riformatrice di un Paese si misura anche dal grado di attenzione che si pone su questioni importanti come questa. La trasmissione di valori positivi e duraturi, come quello della tutela e della valorizzazione del nostro territorio, deve diventare elemento imprescindibile nell'azione di indirizzo e di governo, che partendo dal Parlamento arrivi al livello di ogni amministrazione locale. Il Partito Democratico sostiene convintamente l'ordine del giorno G1. Vorrei ricordare ai colleghi senatori che esso è stato firmato dal Partito Democratico, dal Popolo della Libertà, da SEL, da GAL, dagli autonomisti e dal Partito Socialista Italiano, e da Scelta Civica. A me dispiace che il Movimento 5 Stelle non abbia sottoscritto questo ordine del giorno

c'è bisogno di risorse economiche certe. Bene le riforme costituzionali; bene le riforme di carattere economico sociale. A tutto questo bisogna aggiungere anche la cura e la valorizzazione di questo straordinario, unico - oserei dire - giacimento di bellezza che è il territorio italiano. Il patrimonio paesistico ambientale, storico e culturale non deve essere vissuto come un fardello imbarazzante, ma come una vera e propria opportunità. per ritornare a crescere con stili di vita più appropriati, non meno decorosi, ma sicuramente più responsabili e che, soprattutto, cerchino di lasciare impronte più profonde e positive per le future generazioni.

Ebbene, Presidente, sono rimasto abbastanza sbalordito nel non vedere oggi calendarizzato quel disegno di legge, che avrebbe eventualmente consentito, proprio perché il Governo aveva accolto l'ordine del giorno

Signor Presidente, le chiedo un po' di silenzio e di attenzione da parte dell'Aula: diversamente, credo sia anche inutile intervenire. Colleghi senatori, il Gruppo della Lega Nord ha presentato questa mozione alla luce della necessità di un intervento forte, deciso, ma soprattutto urgente, perché questo fenomeno distruttivo che corre sotto il nome di ludopatia, ovvero dipendenza dal gioco, venga

L'attuale congiuntura economica, superiore per intensità, durata e diffusione a quella del 1929, ha imposto al nostro Paese una politica di contenimento mirata al risanamento dei conti pubblici, con un evidente effetto depressivo e recessivo, tanto da generare un diffuso diffuso impoverimento della cittadinanza e conseguentemente delle famiglie. In un momento difficile come quello che questo Paese sta attraversando (ma forse - ripeto - a nessuno interessa, visto il brusìo) è dovere del Governo tutelare quel sistema di garanzia che si fonda sui rispetto dei principi e dei valori di un Paese civile. I sacrifici richiesti ai cittadini devono trovare risposta negli investimenti costruttivi volti a salvaguardare le strutture fondamentali della società, in primo luogo quindi la famiglia. La famiglia deve tornare ad essere quel valore fondante ed è dovere di questo Governo tutelarne i principi ed i valori stessi. Questa crisi economica ha generato e continua a generare pericolosi fenomeni di carattere sociale: inevitabile assenza di propensione al risparmio ed altrettanto inevitabile ricerca di una ricchezza inesistente; un miraggio e un'illusione, per portare alla definitiva disperazione cittadini e famiglie. Il gioco d'azzardo è ormai considerato la maggior causa di ricorso a debito o ad usura o purtroppo, molto spesso, ad entrambi. Sono ufficiali i dati forniti dalla Consulta nazionale delle fondazioni antiusura, numeri che fanno rabbrividire, come fa rabbrividire sapere che la ludopatia è una delle principali cause di suicidio. I dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono chiari in merito a questo fenomeno, in particolare per quanto riguarda la ripartizione percentuale del gioco d'azzardo: *slot* *machine* 56,7

Su 30 milioni di scommettitori oggi in Italia, ben 15 milioni sono scommettitori abituali e almeno 3 milioni sono a rischio di sviluppare la patologia, senza contare che circa 120.000 già sono dipendenti dal gioco d'azzardo patologico. Ci chiediamo allora come sia possibile che questo Governo neghi l'evidenza di una situazione ormai ingestibile, dovuta alla disperazione e alla fatica del vivere e alle false promesse di un facile arricchimento con vincite inesistenti, perché comunque ‑ ricordiamocelo ‑ vince sempre e solo il banco. La Lega Nord si chiede se questo Governo abbia mai seriamente valutato i costi sociali, diretti ed indiretti, dovuti al danno che questo fenomeno legalizzato comporta: persone annullate, incapaci di smettere, con l'illusione di poterne uscire, dopo aver indebitato le loro famiglie. Uomini e donne, senza distinzione di età o gruppo sociale, che perdono lavoro e dignità, spesso distruggendo anche gli affetti più cari. Persone con le quali l'intervento delle strutture socio‑sanitarie diventa inevitabile; sono: costi sostenuti a fronte di una gestione fallimentare di un fenomeno per il quale la cura può e deve essere una sola: fermare il gioco d'azzardo legato alle *slot* *machine*, valutare attentamente un regolamento, non legalizzare ciò che è vietato dal nostro codice penale. La Lega Nord da sempre, per qualsiasi dipendenza, vede come unica scelta quella del non legalizzare. È come curare la dipendenza dalla droga con il metadone, soluzione da noi sempre contrastata; proibizione drastica e scelta incisiva, dura ma efficace. Non va inoltre sottovalutato l'aspetto della gestione di queste licenze, concesse a società di dubbia natura, a fronte tra l'altro di mancate entrate fiscali che hanno visto premiare evasori, con una sanatoria che ha portato il debito verso l'erario da 98 miliardi a 2,5 miliardi di euro;

onesti ‑ e ripeto la parola: onesti ‑ che con fatica versano il dovuto ad uno Stato che si dimostra iniquo anche sotto questo aspetto. La solita formula: forte con i deboli e debole con i più forti.

è stato introdotto nel Paese il gioco con partecipazione a distanza, vale a dire la licenza, concessa a varie società, per la gestione di apparecchi per il gioco *on line*, con un considerevole aumento del fatturato per le società Non a caso, negli ultimi anni, l'industria del gioco d'azzardo è diventata una delle più importanti del Paese, tanto che *slot machine*, *poker*, scommesse e giochi d'azzardo di diversa natura hanno inondato il mercato a ritmi sempre più frenetici, con notevole crescita del numero dei giocatori, che coinvolge ogni gruppo sociale, compresi pensionati, casalinghe, giovani, e che fa dell'Italia il primo Paese al mondo per spesa *pro capite* dedicata al gioco». mozione quindi: «impegna il Governo a varare in tempi rapidi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti normativi d'urgenza, una moratoria di dodici sul gioco d'azzardo *on line* e sui sistemi di gioco d'azzardo elettronico in luoghi pubblici e aperti al pubblico». Ringrazio chi ha avuto la decenza di ascoltare.

non passa giorno che le cronache non riportino notizie molto spesso drammatiche e dipendenti dalle problematiche del gioco d'azzardo. È certamente un problema atavico, vecchio quanto l'uomo, ma l'opinione pubblica è sempre più preoccupata dalle evidenti correlazioni tra il gioco lecito e quello illecito, ma lo è ancor più di fronte all'impotenza che percepisce nel vedere una continua proliferazione e crescita incontrollata di sale o pseudo tali, in luoghi che non hanno niente a che vedere con l'attività di gioco. Oramai bar, circoli, centri commerciali, sociali, sportivi e ricreati, persino stazioni ed ogni luogo pubblico frequentata diventano occasione di *business*, occasione per piantarci una bella macchinetta (installata sicuramente con tutti i crismi e i protocolli necessari). Migliaia di macchinette che, sembrano essere granelli di sabbia che, uno ad uno, granello su granello, possono trasformare nel tempo un giardino rigoglioso in un deserto. È quel giardino rigoglioso di valori che vogliamo proteggere, qui non si tratta più ormai di difendere posizioni politiche nell'interesse della libera impresa o del libero arbitrio. Anche se il pensiero liberale lascia alla responsabilità di ognuno il compito di regolamentare i servizi che esso eroga o consuma, in questo momento, e anche per gli effetti che ne derivano, non possiamo sottovalutare che il contesto è in continua evoluzione, in particolare quello in cui si sviluppa il gioco d'azzardo illecito. Timidamente il Governo Monti ha parzialmente affrontato il problema con la legge n. 189 del 2012 ma, come ogni legge che si rispetti in questo Paese, l'attuazione è quasi sempre demandata all'emanazione di un decreto volto ad introdurre nuove regole, decreto che per buona pace di tutti, questa volta anche del Governo Letta, è slittato di ulteriori sei mesi. Pazienza, sembrava essere un primo segnale: questo atteso decreto doveva regolamentare espressamente il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, nonché in Internet. Doveva inoltre regolamentare il divieto di ingresso ai minori di diciotto anni nelle sale destinate al gioco con vincite in denaro, nonché mettere mano alla pianificazione ed alla ricollocazione dei locali di raccolta del gioco, anche in relazione alle distanze da scuole di ogni ordine e grado, da strutture sanitarie, di culto, centri socio-ricreativi e sportivi. Pare strano ai più che un tema così importante per i molteplici risvolti etici che ne conseguono, che sono alla base della convivenza civile (pur comprendendo anche quelli di carattere economico, e altrettanto importanti), possa essere regolamentato quasi in via esclusiva dal Ministero dell'economia con il contributo fondamentale dei Monopoli di Stato; ho l'impressione che sia un po' come quel racconto popolare, un po' fantasioso, ispirato ad un noto romanzo di inizio Novecento per cui, anche in presenza di regolari requisiti, il signor Vlad III, conte in Transilvania in tempi addietro, ha rischiato di essere nominato direttore generale dell'AVIS. Per il momento ed in attesa di veder attuate le prime iniziative già approvate si continua comunque a registrare una progressiva esplosione di siti e di pubblicità nelle forme non tutelate e, nel contempo, sta diventando sempre più un'emergenza il fenomeno della ludopatia.

la percentuale di persone tra i quindici e i sessantaquattro anni che ha puntato soldi almeno una volta su uno dei tanti giochi presenti sul mercato è passata dal 42 al 47 si tratta di circa 19 milioni di scommettitori, di cui ben tre milioni a rischio ludopatia, soprattutto uomini, disoccupati e persone con un basso livello di istruzione. Dai dati registrati, emerge la crescita, anche tra gli adolescenti, della febbre del gioco: ammonta a più di un milione il numero di studenti che hanno riferito, nel 2012, di aver puntato denaro sui giochi e, nonostante una chiara legislazione restrittiva a tutela dei minori, risulta che ben 630.000 *under* 18 hanno speso almeno un euro in giochi d'azzardo. Sempre secondo questo studio, un'indagine che ha coinvolto 45.000 studenti delle scuole superiori e 516 istituti scolastici di tutta la Nazione, nell'ultimo anno il 45,3 per cento degli studenti ha puntato somme di denaro. Ad essere maggiormente coinvolti nel gioco risultato essere più i ragazzi che le ragazze e si stima che circa 100.000 studenti già presentino un profilo di rischio moderato e circa 70.000 denotino quelli con una modalità di gioco problematica. Dai recenti dati forniti dai Monopoli di Stato emerge che il settore giochi ha avuto una raccolta di 62.355 milioni di euro nel periodo gennaio-ottobre 2012, con circa 400.000 apparecchi da intrattenimento installati e 6.181 locali o agenzie autorizzate, frequentate da 15 milioni di giocatori abituali. A questo occorre aggiungere che spesso esiste un nesso sempre più stringente tra crisi economica e gioco, che può diventare un potente catalizzatore di malessere e sfiducia. Il mercato del gioco è un settore in costante ascesa e il numero dei malati d'azzardo è destinato pertanto a salire in proporzione al fatturato, alla varietà dell'offerta e all'attrattività del gioco. Ciò che maggiormente preoccupa è che si è di fronte ad una nuova malattia sociale, che sovente genera fenomeni di disgregazione familiare e di impoverimento totale, oltre ad un aumento esponenziale del rischio di cadere nel gravissimo fenomeno dell'usura e della dipendenza. Il gioco sta diventando sempre più una vera e propria illusione di guadagno facile per molte famiglie che si indebitano a causa della dipendenza, e purtroppo molti giovani e ragazzi arrivano a riservare molta più fiducia e speranza nei giochi che nelle istituzioni. Nel nostro Paese, analogamente a quanto succede in altri Paesi dell'Occidente, l'offerta di gioco d'azzardo è in continuo aumento ed è sempre più diversificata, tanto che quella che in passato era un'abitudine riguardante una ristretta fascia di persone è divenuta, di fatto, alla portata di tutti. L'articolo pubblicato su «Avvenire» il 13 giugno scorso riporta dati preoccupanti elaborati dalla Consulta nazionale delle fondazioni e associazioni antiusura, in base ai quali la dedizione ossessiva a *slot machine*, *videopoker* e gratta e vinci sottrae ogni anno 70 milioni di ore lavorative e dirotta almeno 20 miliardi di euro dall'economia reale, cancellando così 115.000 posti di lavoro. È una vera e propria emorragia economica quella provocata dall'azzardo: ne è la prova il tempo usato dai giocatori per le diverse tipologie di gioco. Le nuove *slot machine* hanno totalizzato 28 miliardi di giocate, pari ad oltre 46 milioni di ore passate a schiacciare tasti;

In sostanza, centinaia di milioni di ore perse inseguendo un miraggio. Inoltre, l'azzardo drena risorse ai consumi, già in forte contrazione: se nel 2012 sono stati 90 i miliardi giocati, tenendo conto delle vincite, sono almeno 20 i miliardi di euro sottratti al commercio ed ai servizi destinati alla vendita. Lo studio ha anche calcolato il potenziale di occupazione dissipato dalla spesa per giochi, valutabile in circa 90.000 addetti nel commercio e servizi e circa 25.000 addetti nell'industria. Mi chiedo come si possa, in coscienza, di fronte a questi numeri, assistere quotidianamente alla disgregazione sociale di centinaia di migliaia di famiglie cadute in questa trappola infernale. Non si può rimanere sordi e non capire quale sarà il destino di queste famiglie che, oltre ai beni materiali, perderanno tutto: la dignità, l'onore, il rispetto e la fiducia (la fiducia in se stessi, prima, e nel prossimo, poi). Dietro a questo fenomeno ci sono uomini, donne, anziani e - soprattutto - bambini in carne ed ossa che soffrono e non trovano nemmeno nello Stato quella figura di padre e di nonno che certamente cercano e purtroppo non trovano. Occorrono mezzi adeguati perché, nel più breve tempo possibile, possano essere approvate ed attuate le disposizioni necessarie per evitare che il fenomeno della ludopatia aumenti: ce lo chiedono il buon senso ma anche, con forza, gli organi di stampa, le associazioni di volontariato e gli enti che operano quotidianamente per fronteggiare tali forme di dipendenza. Carissimo Ministero dell'economia, batti un colpo, possibilmente subito e presto! mi avvio a concludere, con l'approvazione di questa mozione in primo luogo si vuole impegnare il Governo ad adottare ogni immediata e tempestiva iniziativa volta ad attuare puntualmente i principi e gli impegni assunti nella XVI legislatura con la conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, al fine di rendere più efficace e incisiva l'azione di contrasto alla ludopatia; 2) ad assumere ogni utile iniziativa volta ad una maggiore tutela dei giocatori, in particolare dei minori e delle altre persone vulnerabili o potenzialmente tali, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da parte dei minorenni; vigilando gli ingressi e formando *ad hoc* il personale, nonché vigilando in pari modo sul gioco *on line*; attraverso campagne informative di prevenzione; a proseguire nella promozione di iniziative di sensibilizzazione circa i rischi collegati al gioco e di azioni restrittive, oltre che di controllo e monitoraggio, dirette ad arginare il fenomeno del gioco, soprattutto ad opera dei minorenni più facilmente condizionabili e suscettibili, e nei quali la tendenza alla dipendenza è molto più alta.

premesso che: nel corso degli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto un volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Purtroppo, è ormai evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie forme di scommesse, lotterie e apparecchi elettronici,

nonché il gioco clandestino, con un volume di spesa che ha raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 164 miliardi di euro negli ultimi 6 anni; il gioco d'azzardo sta diventando una vera e propria emergenza sociale, soprattutto alla luce del fatto che i maggiori giocatori sono i giovani, di pari passo con la diffusione del gioco d'azzardo si ha una preoccupante diffusione della ludopatia (definita GAP, gioco d'azzardo patologico). Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo psichiatrico classificato come un disturbo del controllo degli impulsi ed è caratterizzato da una sintomatologia ossessivo-compulsiva. Esso è un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette dipendenze da sostanze. Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco; tra le conseguenze più evidenti provocate da tale patologia vi sono sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi; a ciò si aggiungano i rischi di associazioni ad altre dipendenze, soprattutto alcool e stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo *stress*. Attualmente tale patologia sta iniziando a colpire sempre più i giovani, a causa della facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. Si consideri, inoltre, che la gravità della situazione si può riscontrare anche nel fatto che che i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologico sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione. Una realtà, quella descritta, che non può passare inosservata. In effetti, anche in considerazione della necessità di contrasto e prevenzione della ludopatia, il gioco d'azzardo negli ultimi decenni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a disciplinare l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;

che le amministrazioni, nell'esercizio dei rispettivi poteri, devono agire nel rispetto delle prescrizioni di legge volte a stabilire i requisiti dei locali adibiti a sale giochi, tutelando il diritto costituzionalmente garantito alla salute, provvedendo ad annullare, revocare e disporre i controlli necessari per garantire il rispetto dei divieti di pubblicità e gioco ai minori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle VLT; all'art. 1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

189 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia,

preso atto che il "decreto Balduzzi" ha previsto inoltre l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita nelle aree e nelle sale con videoterminali, e ha dettato nuove regole in tema di pubblicità dei giochi; le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti debbano essere rilasciate in presenza di adeguata istruttoria e puntualmente motivate in sede di giustificazione del loro rilascio, impegna il Governo: 1) ad utilizzare strumenti e procedure concrete per verificare sul territorio che le autorizzazioni rilasciate per l'installazione delle VLT rispettino la normativa a valutare proposte ovvero iniziative volte a stabilire protocolli di sicurezza oltre a quelli attualmente previsti; 3) a contrastare il fenomeno del GAP legato alle VLT considerata l'evidente urgenza di regolamentazione del fenomeno e considerato altresì che il ritardo nell'adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quanto fino ad oggi realizzato rappresenta un grave lacuna e un preoccupante stallo nella prevenzione della ludopatia; ad adottare una strategia ed iniziative per rendere operativi i principi contenuti nel decreto Balduzzi, anche con riferimento ai finanziamenti dedicati e finalizzati all'avvio sistematico di iniziative di cura e prevenzione per contrastare il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo; a proporre un preciso limite al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione nelle sale da gioco delle VLT; 6) a prevedere una organica disciplina *ad hoc* per le VLT che tuteli i soggetti a rischio ludopatia.

declino, di un Paese che non riesce ancora a fare della crisi una risorsa potente per cambiare e fare leva su un binomio inedito e virtuoso di legalità e sviluppo; gioco d'azzardo e compra-oro sono invece un circolo vizioso che rende il nostro Paese dipendente e ricattato dai suoi stessi limiti strutturali. Presidente, nel gioco d'azzardo il fatturato si aggira intorno ai 90 miliardi di euro, una cifra pari al 4 per cento del PIL nazionale. Se volessimo fare un paragone con le grandi imprese del nostro Paese, collocheremmo il fatturato del gioco d'azzardo SpA al terzo posto dopo l'ENI e l'ENEL. Nello stesso tempo - ecco qui il paradosso

ci troviamo, a fronte di una fatturato enorme, smisurato, un incasso piccolo; ma quel piccolo incasso di 9 miliardi di euro è indispensabile per la tenuta dei nostri conti. Di qui il ricatto, il limite strutturale: un circolo vizioso. Di recente abbiamo avuto un *report*, realizzato da Avviso Pubblico, quella realtà che associa enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, che ci ha spiegato bene come si esercita questo ricatto, i danni che subisce il nostro Paese, gli effetti collaterali che si scaricano sulle persone dipendenti che partecipano al gioco d'azzardo. Ecco perché giocatori di 30 milioni di persone, di cui 2 milioni a rischio dipendenza e 800.000 giocatori patologici, una cifra doppia a quella dei tossicodipendenti presenti in Italia.

con enormi carenze di personale e poche risorse, ad intervenire su questa nuova sfida che sta mettendo in seria difficoltà giovani, persone adulte e famiglie del nostro Paese. Paese. Anche la facilità di accesso ai giochi d'azzardo e l'enorme presenza di pubblicità sui mezzi di informazione e comunicazione, spesso anche con formule ingannevoli, contribuiscono ad aumentare il rischio. *Slogan* come «Ti piace vincere facile»

nei livelli essenziali di assistenza, cosa che è avvenuta dopo trent'anni, quindi «con un po' di ritardo». Il decreto Balduzzi di qualche mese fa ha introdotto la dipendenza dai giochi nei LEA, cioè nei livelli assistenziali, ed entro poco tempo (il 31 dicembre 2012), su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovuto provvedere ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 si prevedeva inoltre il divieto d'ingresso per i minorenni nelle aree destinate al gioco con vincite di denaro interne alle sale Bingo, nonché alle aree in cui si installano i videoterminali e nei punti vendita dove si esercita come attività principale quella di scommessa. Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, non sono stati adottati né il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'aggiornamento dei livelli di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione, né il suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sul divieto relativo ai minori. Ecco perché c'è un limite strutturale, ecco perché questo ricatto strisciante pesa sulla vita democratica ed economica del nostro Paese. In passato questo Parlamento si è occupato del gioco d'azzardo, ha denunciato il vuoto enorme che c'è, in particolare sul gioco d'azzardo *online*, terra di nessuno, di arricchimenti spropositati, di dipendenza, di presenza delle mafie, di introiti stupidi, bassissimi e di controllo di legalità pari a zero. Eppure, il Parlamento si è pronunciato nella passata legislatura più volte: ricordo interventi di autorevoli nostri parlamentari, che oggi non siedono più in Aula e che si sono battuti intorno alla

ecco perché il Partito Democratico ha presentato una mozione dettagliata con la quale si chiedono impegni seri, seri, si invita il Governo ad assumersi delle responsabilità certe, e a fare i conti con la presenza delle organizzazioni mafiose, ricordando che queste hanno raggiunto un fatturato di circa 10 miliardi di euro. Sono presenti tutte le organizzazioni mafiose (cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita). Attorno a questo grande affare, l'associazione Libera ha censito la presenza di ben 50 clan con interessi diretti e indiretti: ricordiamo i casalesi, i Santapaola, i Condello, i Lo Piccolo: e l'elenco sarebbe lungo da fare. Per questo, cari colleghi, abbiamo pensato di proporre una mozione ben dettagliata. Ecco perché, colleghi, invitiamo il Governo - e invito il rappresentante del Governo a prenderne nota

di chiudere il contenzioso aperto con i concessionari di giochi pubblici per il mancato versamento di quanto dovuto all'Erario, garantendo un'entrata certa in tempi ravvicinati, chiudendo così procedimenti aperti da anni, ma - attenzione - dove erano in gioco miliardi e miliardi di euro che i concessionari devono allo Stato. Penso che questa copertura debba essere rivista; penso che in Parlamento ci dobbiamo impegnare insieme al Governo per evitare che ancora una volta i giochi d'azzardo siano considerati una risorsa: sono un limite, sono un problema, sono un ostacolo allo sviluppo e alla legalità del nostro Paese. Nei nostri impegni individuiamo la necessità di elevare gli *standard* di accreditamento dei concessionari e il sistema dei controlli sulla loro identità societaria, sull'origine dei loro patrimoni e sui loro flussi finanziari attraverso un sistema di tracciamento dei movimenti in entrata e in uscita, al fine di evitare la presenza di infiltrazioni mafiose e di riciclaggio di denaro sporco. ad introdurre, per quanto riguarda la tracciabilità del denaro, il conto dedicato e il registro delle scommesse e dei concorsi pronostici; ad introdurre il divieto di partecipare a gare e procedure per il rilascio di concessioni in materia di giochi da parte delle persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi; a stabilire per società fiduciarie, fondi di investimento e *trust* che detengono partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante; ad equiparare agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in Italia senza licenza; ad istituire presso tutte le procure della Repubblica

da questo affare lo Stato subisce perdite miliardarie. Terzo: è un terreno di coltura per illegalità e fenomeni mafiosi. Quattro le nostre proposte di soluzione, quelle che il Paese chiede. Non è un gioco, ma un comportamento rischioso per la salute. I giocatori in Italia sono circa 15 milioni, di cui 1.250.000 sono ragazzi tra i quindici e i Le stime più restrittive calcolano in 800.000 i giocatori patologici e in 2 milioni i giocatori problematici; gli adolescenti tra i 15 e i 19 anni, con profili di gioco problematico o patologico, secondo le recenti indagini pubblicate dal Dipartimento delle politiche antidroga, sono il 7,2 per cento, cioè circa 200.000. Il gioco sarebbe vietato ai minorenni: hanno un sistema emotivo in fase di sviluppo e un minore controllo degli impulsi, sono dunque più vulnerabili e vanno protetti. La varietà, la disponibilità e l'accessibilità dei giochi, invece, facilitano l'insorgenza della patologia, come pure la pubblicità, specialmente quella ingannevole, e, ancora, il breve tempo di latenza tra la giocata e il suo esito, che nelle *slot machine* è di qualche secondo appena. Il gioco d'azzardo patologico è molto simile alla dipendenza da droghe. Il desiderio irresistibile porta a trascurare il lavoro, gli affetti, la famiglia, i figli, a commettere reati o a restarne vittima, come nel caso dell'usura. sanitario nazionale non ha ancora istituito programmi di prevenzione e cura. Si è previsto l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, ma non ci sono coperture economiche e dunque in Conferenza unificata Stato-Regioni non si è dato seguito ai proclami.

ad una tassazione media del 9 per cento. La sola IVA per le nostre imprese è invece attualmente al 21 per cento. È una disparità inaccettabile, un favore troppo eclatante per non risultare sospetto. Questo fatturato deriva per il 56 per cento da *slot machine* e *videolottery*, che pochi anni fa non esistevano, e buona parte del mercato è in mano a multinazionali residenti in paradisi fiscali.

Lo Stato da parte sua perde, per mancati consumi, circa 3,8 miliardi di entrate IVA. L'attrazione per il gioco causa poi assenteismo. È correlata a patologie da *stress*, a problemi psicologici anche gravi (ansia, depressioni, idee suicidarie) e a dipendenza da alcol e droghe. I giocatori patologici richiedono dunque più assistenza ambulatoriale e ricoveri, hanno maggiori assenze per malattia, denotano minore produttività sui luoghi di lavoro e, spesso, lo perdono, il lavoro. Dunque le famiglie necessitano di assistenza sociale. Consideriamo poi i danni derivanti da furti, truffe, usura e i costi per lo Stato per il contrasto ai fenomeni criminosi. i costi sociali e sanitari per l'Italia ammonterebbero a circa 6 miliardi. Dunque l'Italia ricava 8 miliardi l'anno, ma le entrate per l'Erario sono in calo, mentre subisce perdite per 10 miliardi e le patologie sono in aumento. A chi conviene questo mercato? Vengo al terzo punto. Il mercato illegale vale 10 miliardi. Almeno 42 cosche, qualcuno dice 50, a seconda dei conteggi, probabilmente sono di più, sono state indagate da dieci procure per gli interessi anche nel mercato legale, che vale 88,5 miliardi nel 2012 e viene utilizzato come lavanderia per riciclare capitali sporchi, poiché i flussi di denaro non vengono adeguatamente monitorati. Nemmeno il divieto del gioco per minorenni viene fatto rispettare. La Commissione parlamentare antimafia nella scorsa legislatura ha denunciato i gravi fenomeni di illegalità legati al settore: usura, estorsioni, riciclaggio di denaro, truffe, elusione ed evasione. Grosse responsabilità ha la politica, che a partire dal 1997, da destra a sinistra, ha di fatto rovesciato la normativa: ciò che prima per legge era vietato, con poche eccezioni, è diventato usuale. L'eccezione ha ucciso la norma. Quarto punto. Quali misure devono essere adottate? *In primis* attribuire maggiori poteri ai sindaci per regolare la diffusione dei locali e la loro attività. La normativa attribuisce questa responsabilità alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, estromettendo i sindaci dai compiti di tutela della salute pubblica. istituire un registro nazionale per le persone che, per proteggersi, chiedono volontariamente di essere escluse dall'accesso ai giochi, come già avviene nei casinò, ed introdurre sistemi di accertamento dell'identità anche a tutela dei minori.

Il decreto-legge n. 158 del 2012 impone che sugli apparecchi elettronici e negli spazi adibiti al gioco d'azzardo siano visibili avvertenze sui rischi. Deve essere tuttavia spiegato

«evidente». Le vincite, il cui ammontare sia pressoché pari alla giocata, non devono essere considerate nel computo: se cioè metto un euro e ricevo un euro, dov'è la vincita? Il giocatore ha però una falsa sensazione di gratificazione, che lo incentiva al gioco. Con questo sistema, inoltre, la probabilità di vincita viene artificialmente gonfiata. È necessario allineare ed uniformare la tassazione sui diversi giochi, innalzandola già a partire dall'anno in corso. Le maggiori entrate devono essere destinate al finanziamento di programmi di prevenzione, cura e ricerca e dare, quindi, piena applicazione al decreto-legge n. 158 del 2012. si finanzi, di concerto con le associazioni promotrici della campagna nazionale contro i rischi da gioco d'azzardo «Mettiamoci in gioco», uno studio che determini quanto costerebbe e quali benefici potremmo trarre dal ritorno alla situazione normativa antecedente al 1997, quando non avevamo *slot machine* e vivevamo meglio,

incrementare le sanzioni penali ed amministrative per coloro che esercitano, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse in mancanza di autorizzazione o licenza; assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari nel gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, per prevenire infiltrazioni criminali e riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Infine, bisognerebbe promuovere nel corso dell'esame parlamentare del cosiddetto decreto IMU la soppressione dell'articolo 14, attivando le procedure necessarie per esigere integralmente le somme dovute dalle imprese operanti nel settore del gioco d'azzardo fiscale *(Applausi dal Gruppo M5S)* e rimuovere immediatamente da ruoli di responsabilità e di discrezionalità i funzionari dello Stato coinvolti a vario titolo in questa scandalosa vicenda giudiziaria.

Signor Presidente, l'argomento che ci troviamo ad affrontare oggi è di particolare rilievo sociale, vista e considerata la diretta correlazione tra l'espansione del mercato del gioco e l'incremento dei cosiddetti malati di azzardo. La febbre da gioco è identificabile come una vera patologia, con una chiara sintomatologia. L'*input* iniziale è spesso la ricerca di emozioni forti e di facili guadagni, del colpo di fortuna che spinge a tentare la carta del gioco, magari credendo di sperimentare una nuova evasione, quando in realtà si cade nel vortice di quello che diventa un vero e proprio vizio, un incontrollabile impulso caratterizzato dall'alternanza di fasi di depressione e di euforia. Ciò che risulta più allarmante è la mancanza di consapevolezza dei rischi che si corrono quando ci si lascia ammaliare dal gioco. Le campagne di *marketing* pubblicitario che promuovono l'industria dei giochi d'azzardo sui *media* esaltano i facili guadagni e sono di gran lunga più diffuse rispetto alle campagne che invece dovrebbero, responsabilmente, gettare luce sulle componenti psicologiche e sociali legate al fenomeno, alla possibilità di perdere il controllo e alla cognizione dei limiti oltre i quali non bisogna spingersi. Si parla tanto degli effetti nocivi del fumo, delle sostanze stupefacenti e dell'alcol, ricorrendo ad immagini forti per demotivarne l'uso: le campagne di prevenzione in questi casi sono numerose ed anche piuttosto efficaci. Certamente un passo avanti si è fatto con la legge n. 189 del 2012 che, tra le altre cose, ha giustamente previsto il divieto di pubblicità di pubblicità che inducano al gioco su riviste, quotidiani, nei cinema e su Internet. Le cifre parlano chiaro e riportano statistiche allarmanti, come hanno detto bene coloro che hanno illustrato le mozioni. Si parla di 30 milioni di scommettitori nel nostro Paese, di cui 15 milioni abituali e almeno 3 milioni a rischio di sviluppare una patologia. Il dato più preoccupante in assoluto, però, è che questo numero è in continua crescita proprio tra le fasce più deboli della nostra società, tra coloro che non hanno ancora gli strumenti adeguati per valutare rischi e ripercussioni, e sono quindi maggiormente soggetti a sviluppare una dipendenza, come gli adolescenti. Per questo è necessario introdurre misure ancora più restrittive all'accesso alle aree destinate al gioco e alle scommesse, a tutela dei minori, e diffondere campagne informative anche nelle scuole, con successive azioni di monitoraggio e controllo fra i più giovani. Fra gli aspetti più rilevanti di un'efficace strategia di prevenzione, va evidenziata l'esigenza di collocare, come prevede la legge, i punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante apparecchi elettronici lontano dalle zone sensibili, come gli istituti di istruzione primaria e secondaria, le strutture sanitarie e ospedaliere, i luoghi di culto e i centri socio ricreativi e sportivi. Su questo punto è necessario emanare presto i regolamenti attuativi, poi sarà necessario un serio controllo per contrastare efficacemente eventuali violazioni. Inoltre, la febbre da gioco è diventata una vera e propria patologia sociale con implicazioni e risvolti che toccano la sfera psicologica, economica, affettiva e lavorativa. Proprio per contrastare il fenomeno alla sua radice, un'adeguata campagna sociale di sensibilizzazione ed informazione può contrapporsi all'illusione di guadagni facili. Il messaggio distorto che viene ancora trasmesso, soprattutto fra i più giovani, è quello di un gioco d'azzardo come formula di guadagno facile ed immediato, che non richiede nessun tipo di impegno: una sorta di comoda alternativa ad investire tempo ed energie nello studio Soprattutto in una fase congiunturale critica, in cui si è ancor più vulnerabili alla tentazione di prospettive di guadagno facile, dovremmo intervenire in maniera energica per contrastare questo falso mito. Nonostante le entrate derivanti dal gioco d'azzardo siano elevate, in una valutazione del rapporto costi-benefici che tenga conto degli effetti sociali ed economici generati da un'ulteriore espansione dell'industria del gioco nel Paese, non solo emerge la preoccupazione per questa nuova forma di patologia sociale, la ludopatia, ma si evidenziano anche conseguenze economiche tutt'altro che trascurabili. L'azzardo drena infatti risorse ai consumi, che già risultano in forte contrazione, determinando una vera e propria emorragia economica, e ruba inoltre un'altra risorsa dal valore inestimabile al mercato del lavoro, il tempo. Sarebbero quindi necessarie e auspicabili misure restrittive per scoraggiare l'accesso dei più giovani al mondo del gioco d'azzardo per regolamentare in maniera più rigida il suo funzionamento con forme di controllo stringate e capillari, valutando anche la possibilità di fissare limiti massimi consentiti per le somme da per le somme da giocare. Laddove si rischia di mettere a repentaglio il benessere dei nostri giovani, non c'è partita che tenga, ed i costi sociali sono di gran lunga più elevati di quelli rappresentati dalle entrate... *(Il microfono

Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho sempre appoggiato qualsiasi iniziativa che porti ad una restrizione e ad un maggiore controllo di ciò che si sta delineando, non solo in Italia ma in tutta Europa, una piaga terribile: il gioco d'azzardo. Leggendo tutte le motivazioni che sono state apportate nelle mozioni che andremo a votare, questa si concentrano sulle problematiche sociali che il gioco d'azzardo innesca attraverso la sua forma la sua forma più grave, la ludopatia, a tutti i livelli della società, che coinvolge una ampia fascia di popolazione, soprattutto minorenni, giovani e anziani che non si possono difendere nel modo più adeguato. Tutte motivazioni veritiere nella loro drammaticità, che comportano oltre alla dilapidazione di interi patrimoni familiari, l'indebitamento estremo che spinge nel gravissimo fenomeno dell'usura le persone che già si trovano in difficoltà, sino all'atto estremo dei suicidi per debiti dei giocatori stessi. Quello che secondo me mettono chiaramente in luce sono le conseguenze, ma non le cause, non spiegano chi si arricchisce e alimenta questo fenomeno. Sto parlando della criminalità, che si sta trovando spazi, territori da controllare, proprio con il gioco d'azzardo e le attività illecite ad esso collegate, si sta insinuando in territori sempre più vasti dell'Italia e lo Stato non deve assolutamente cedere. Le organizzazioni malavitose utilizzano questo mezzo, le sale gioco e il gioco d'azzardo, per riciclare il denaro che ha una provenienza illecita e per rubare l'innocenza di tanti ragazzi che per ingenuità o curiosità si avvicinano a queste sale. Quindi studiare ulteriori strumenti normativi che mettano un freno a questo fenomeno, che aumentino i controlli e l'inasprimento di tutto quello che è l'*iter* burocratico per l'apertura di queste sale è sempre di buon auspicio. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, arrivo da una Provincia, quella di Imperia, che è famosa perché ha come simbolo la città di Sanremo e il suo casinò comunale, che attua un rigido controllo a chi entra e all'età delle persone che ne usufruiscono. Proprio per questo controllo, oggi si trova sull'orlo del fallimento. Inoltre proprio la diffusione che ha il gioco d'azzardo da parte della criminalità organizzata sta portando a ulteriori conseguenze che a prima vista non sembrano collegate. Quelle amministrazioni o singoli amministratori che si oppongono all'apertura di nuove sale da gioco sono minacciati di morte. Questo lo so perché io sono una di quegli amministratori, mi sono opposta con tutte le mie forze all'apertura di un'ulteriore sala da gioco nel mio Comune, ho avuto il coraggio di denunciare e per questo motivo ho vissuto un anno e mezzo sotto scorta. Il periodo più difficile e travagliato della mia vita, ma lo rifarei senza indugi per difendere la comunità a cui appartengo. Anche per questa motivazione, trovo importante che lo Stato sia presente, in questo territorio,

Signor Presidente, intervengo brevemente, anche perché le mozioni che sono state illustrate sono pienamente condivisibili. La lotta alle ludopatie rappresenta sicuramente un'importante sfida per la società e in particolare per il nostro sistema sanitario, quindi condivido in pieno le considerazioni e gli impegni che tali mozioni contengono.

aspetto a dir poco preoccupante, che potrà essere combattuto solo con un reale impegno da parte delle stesse famiglie volto a indirizzare i propri figli ad attività umanizzanti e formative, come la musica e lo sport, in luogo di usare in modo comodo e semplice le TV o i computer come nuovi *babysitter*. Vorrei però sottolineare un aspetto particolare,

riconosciuti. Ricordo che le quattro case da gioco autorizzate (Campione d'Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia) promuovono una cultura del gioco consapevole e responsabile: hanno infatti tutte stipulato una convenzione con aziende sanitarie di riferimento e con dipartimenti di salute mentale, nell'ottica di una politica legata alla prevenzione dei rischi relativi alla dipendenza da gioco d'azzardo. Esiste ad esempio la possibilità di richiedere l'autoesclusione o la limitazione da parte dei giocatori stessi o delle loro famiglie dalle case da gioco, cosa invece improponibile e impensabile nelle forme di gioco come il Superenalotto, il *poker online* e così e così via. L'aumento dei casi di ludopatia è legato soprattutto alle forme di gioco al di fuori dei casinò autorizzati, che hanno visto invece una drastica riduzione di clienti. Quindi, le iniziative legate al rilancio dei casinò, come l'innalzamento del limite del contante, hanno non solo la finalità di cercare di risollevare le sorti di un settore in crisi, che coinvolge più più di 3.000 dipendenti, ma anche quella di fare ridiventare le case da gioco e i casinò strutture privilegiate per chi vuole giocare in modo controllato e sicuro, dove - lo ricordo - tutto il denaro è tracciato

una sorta di ossimoro concettuale, possiamo dire, o di tipo contenutistico. Certo, i dati relativi al gioco d'azzardo indotto sono impressionanti. Non più tardi del luglio 2012, l'agenzia britannica Reuters affermava che, anche in un momento di profonda crisi economica, la promessa di un *jackpot* in Italia brilla ad ogni angolo di strada l'Italia è il più grande mercato del gioco d'azzardo in Europa e uno dei più grandi al mondo. Secondo la Consulta nazionale antiusura e le fondazioni antiusura, il gioco d'azzardo è considerato la maggior causa di ricorso a debiti e/o di usura in Italia.

percorsi che lentamente ed inesorabilmente conducono allo smarrimento, all'isolamento sociale ed affettivo, all'indebitamento, al ricorso ad illegalità ancor più ampie e distruttive. La morte del ragazzo è solo l'ultima prova di un'emergenza che è scoppiata in Italia. Ormai, il rischio di sviluppare forme di dipendenza dal gioco si è esteso ai più giovani: una dipendenza ancor più pericolosa, perché si sviluppa dentro casa, nell'intimità familiare potremmo dire, giocando e perdendo soldi davanti ad un computer, utilizzando Internet. Siamo testimoni di una subdola e pervadente emergenza e deriva sociale, che deve essere assolutamente contrastata, adottando misure atte a difendere soprattutto i più giovani, e non solo loro, direi. Ben vengano mozioni ed iniziative varie volte a contrastare ed emarginare il fenomeno, ma il tema in oggetto è di una tale gravità sociale che non possiamo ritenere di limitarlo con la sola forza delle mozioni. Dobbiamo andare oltre. Gioco d'azzardo e ludopatie sono questioni strutturali, che interpellano noi tutti e richiedono lo sviluppo e la realizzazione di politiche che siano davvero e coerentemente orientate alla tutela di ogni persona, della sua dignità, dei nuclei familiari, al contrasto del fenomeno. Insomma, diciamolo chiaramente e con forza, questa sera: non si possono liberalizzare i giochi d'azzardo alla ricerca di entrate fiscali per lo Stato

quando, per già evidenti ragioni economiche, l'Italia aveva bisogno urgente di entrate fiscali. Nel 1994, il fatturato non superava comunque i 6,5 miliardi di lire. Qualcuno, a questo punto, potrebbe obiettare e dire che si tratta di realismo politico: in ragione di un'economia dello Stato, è possibile fare anche questo.

Poco più tardi, nel 2011, con il cosiddetto decreto di Ferragosto, è stata avviata la liberalizzazione dei giochi d'azzardo *online*. Il fatturato del gioco *online* è solo una parte di quello del gioco d'azzardo nel suo insieme ed è anche il settore che è cresciuto di più, con un aumento, rispetto al 2011, del 100 per cento. Nei primi sei mesi, dopo la liberalizzazione, sono stati fatturati più di 5 miliardi di euro.

Diceva Hemingway in un suo famoso scritto: se suona la campana, quella campana suona anche per te.

Anche oggi, grazie all'impulso fornito dalle mozioni presentate dai colleghi, intendiamo chiedere al Governo un impegno serio su come affrontare questo delicato problema. ormai risaputo che il gioco d'azzardo è diventato un'attività che comporta pesantissimi e notevoli rischi per la salute e non solo per quest'ultima. Lo sappiamo tutti che il gioco d'azzardo è una piaga sociale che sta influenzando l'economia nazionale, quale disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette dipendenze senza sostanze. Nel giocatore si denota una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, poiché egli aumenta la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare e la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investe più delle proprie possibilità economiche e trascura i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco. Bingo, Gratta e vinci, giocate al Lotto o al Superenalotto, *slot machines*, *skill games*, scommesse di ogni genere, legali e non, sono fattori che stanno accentuando il passaggio dal gioco consapevole e controllato al dramma del gioco d'azzardo patologico. Su diversi aspetti preoccupanti della nostra società, spesso ricollegabili alla crisi economica, è stato avviato un monitoraggio dei riflessi sul piano della sicurezza del fenomeno della ludopatia, negli ambiti di intervento della direttiva sul disagio sociale che il Ministero dell'interno ha inviato a tutte le prefetture. Il testo, che punta a prevenire le possibili tensioni sui territori generate dalla crisi economica, è stato presentato alla stampa lo scorso 9 luglio dal capo di gabinetto del Ministero, Giuseppe Procaccini. uno studio dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa, sarebbero più di un milione gli studenti che lo scorso anno avrebbero riferito di aver giocato del denaro e, nonostante una chiara legislazione restrittiva per i minori, anche 630.000 *under* 18 hanno scommesso almeno un euro. Siamo tutti al corrente del fatto che l'allarme sociale riguarda soprattutto gli uomini, i disoccupati e le persone con un basso livello di istruzione, ma non è vero: la platea dei giocatori non fa altro che allargarsi, sino a comprendere padri in cassa integrazione, giovani, pensionati e perfino casalinghe. Saremmo degli ipocriti se chiudessimo gli occhi: forse perché vanno tutelati gli interessi delle solite potenti *lobby* che condizionano l'azione politica del Governo in materia di gioco d'azzardo? Non si può accettare né tanto meno permettere che in Italia si faccia, con sotterfugi che ormai tutti conosciamo, una campagna di fidelizzazione del giocatore accanito, a discapito della sua salute fisica, morale oltre che della sua dignità. Altrettanto pericoloso è il gioco d'azzardo *online*, in cui il giocatore diventa prigioniero di se stesso nella solitudine di una stanza e di un computer che non viene mai spento. Per aiutare questi soggetti ad uscire dalla dipendenza, nei SERT presso le varie aziende sanitarie provinciali, (ASP) ci sono *équipe* di professionisti, psichiatri, psicologi, assistenti sociali ed educatori che si occupano della diagnosi e della cura che sono oggi ben preparati per la cura delle dipendenze da droghe e alcol, ma non del gioco d'azzardo. A causa dei limitati se non scarsi *budget* stanziati in favore delle singole ASP, purtroppo si assiste sempre più ad una inadeguata risposta da parte di questi servizi, vuoi per carenza di personale, vuoi per mancanza di formazione e aggiornamento *dell'équipe* medica, ma soprattutto per carenza di luoghi dove sia possibile curare in maniera riservata. Non è inutile evidenziare che il soggetto affetto da GAP (gioco d'azzardo patologico) prova vergogna a dichiarare la sua patologia, ma soprattutto per *forma mentis* o per formazione culturale non vorrà farsi curare in una struttura dove vengono curati i dipendenti da sostanze stupefacenti. Forse dovremmo chiederci se non è il caso di istituire, presso i dipartimenti per le dipendenze già attivi presso ogni ASP, un'unità operativa competente in materia di patologie riconducibili al gioco d'azzardo patologico, per la presa in carico multidisciplinare dei soggetti affetti da GAP, o predisporre percorsi formativi *ad hoc* sul trattamento delle patologie riconducibili al gioco d'azzardo dedicati agli operatori sociosanitari. Sarebbe opportuno iniziare serie collaborazioni con le istituzioni scolastiche per attività di prevenzione sui minori, così come iniziare campagne di sensibilizzazione volte a fare comprendere che dal *tunnel* del gioco d'azzardo si può uscire anche attraverso il temporaneo riconoscimento dell'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno che tuteli il patrimonio del soggetto affetto da GAP. Il gioco d'azzardo infatti è considerato giorno dopo giorno sempre più, in tempo di crisi, una via di uscita da situazioni di povertà. Soltanto dopo essere caduti nel vortice, però, ci si rende conto di essere finiti nelle grinfie di un mostro che tutto può, tranne che sollevare la propria economia. Contro l'azzardo non si possono non intessere legami a livello nazionale, regionale e perfino comunale: insieme si deve lavorare per vietare l'istituzione di nuovi giochi con vincite in denaro, potenziare gli esistenti centri e servizi di assistenza, creare un fondo per la prevenzione, nonché cura e riabilitazione da gioco d'azzardo, e tutelare i minorenni, ad esempio riducendo i tempi di gioco. Non ci si può esimere dall'individuare le vere responsabilità, ad esempio quelle che dovrebbero attribuirsi a chi propina pubblicità spesso ingannevoli, le quali si rivolgono, come *target,* proprio alle fasce più deboli. parte delle istituzioni dovremmo forse iniziare a pensare di introdurre una tassa a carico dei locali con *slot machine* per finanziare la cura del gioco d'azzardo patologico, e prevedere l'opportunità per i Comuni di regolare gli spazi di gioco all'interno dei locali, a vietare di pubblicizzare il gioco d'azzardo, prevedendo magari incentivi per chi rinuncia alle *slot* *machine* o le toglie dai propri locali. Siamo espressione dello Stato e abbiamo il dovere di rispettare la Costituzione, che ha sancito un diritto chiaro e preciso al primo comma dell'articolo 32: 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il Governo deve impegnarsi ad individuare la linea più efficace per combattere il tarlo del gioco. Non può fare giochetti sporchi anche in quest'occasione: la gente che si ammala si aspetta garanzie, tutele e soprattutto riconoscimento di dignità. Il dramma del gioco d'azzardo è una pagina triste della storia italiana, che pare non si voglia voltare, per quel contraddittorio, se non lurido, rapporto tra la filiera del gioco e la politica speculativa. Non possiamo accettare, soprattutto in un periodo storico come questo, in cui l'economia e le famiglie sono in ginocchio, che il Governo decida di agevolare gli interessi del comparto del gioco. modo, noi del Movimento 5 Stelle non accettiamo la presa di posizione di questo Governo sul megacondono delle sanzioni da applicare ai *boss* dell'azzardo. La questione, invece, è ben più subdola e puzza di marcio. Tutti sappiamo che il Governo Letta, come parziale copertura del decreto-legge sull'IMU, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, ha inserito 600 milioni di euro provenienti da concessionari di *slot machine* su cui pende una multa di 2,5 miliardi. Insomma, attraverso una sanatoria lo Stato chiederebbe alle dieci società multate in primo grado dalla Corte dei conti, che già hanno presentato ricorso in appello, di chiudere le proprie pendenze versando appena un quarto del dovuto. Giusto per non dimenticare i nomi delle società concessionarie multate, le cito velocemente: G.Matica srl, Codere SpA, HBG srl, Gamenet SpA, Cogetech SpA e la famosa SNAI SpA. Si ricorda che il danno erariale stimato è pari a circa 98 miliardi di euro, in conseguenza della ritardata attivazione della rete telematica di controllo. Infatti, a scanso di equivoci, il Governo ha messo le mani avanti esplicitando che, qualora dovesse emergere un andamento che non consentirà il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze sarà tenuto ad aumentare la misura degli acconti ai fini IRES e IRAP e, contestualmente, le accise. Tuttavia, la maggiorazione nei prelievi di IRES e IRAP e un aumento delle accise potranno probabilmente toccare alcol e tabacchi e rimarrebbero salvi i giochi, in quanto soggetti a tassazione ordinaria e non ad accisa. Bello, no? Caro Governo, con tutti i suoi pregevoli Ministri, mi pongo una domanda da parecchio: ma non vi siete stancati di prendere in giro la gente? Soprattutto, riuscite ogni mattina a guardarvi allo specchio, oppure avete smesso di farlo per paura che vi risponda male?

non vi è dubbio che vi siano problemi legati alla legalità e ad un mercato molto complicato e variegato. Tuttavia, con il mio intervento desidero mettere l'accento sulla questione della salute e sul tema drammatico tutela dei minori. *online* sono utilizzati in modo del tutto deregolato dai minori. Questo è un problema che interroga la civiltà di un Parlamento e di un Paese. Non è pensabile,

mentre nelle sale è più semplice vedere i cartelli di divieto, all'interno dell'infinità di bar in cui ci sono le *slot* *machine* è molto difficile vedere cartelli di divieto ai minori. Il problema Il problema si risolve non facendo un proibizionismo *d'antan*, ma coinvolgendo i diversi attori del problema, tra i quali vi sono anche i produttori di giochi e gli esercenti. È inutile che continuiamo a predicare un ruolo della scuola e della famiglia

Vorrei che non usassimo più il termine ludopatia perché è sbagliato. Quando c'è la dipendenza da gioco d'azzardo, che è una patologia specifica, bisogna che il nostro Stato la riconosca, e attualmente non è così, perché non è presente nei livelli essenziali di assistenza, a dispetto di quanto è stato detto dall'Organizzazione mondiale della sanità e dai trattati internazionali che la definiscono una patologia pari

C'è un servizio specifico - ne parlava la collega prima - che si chiama SERT; c'è una federazione italiana che si chiama Federserd, che riunisce tutti coloro che si occupano delle patologie legate al gioco d'azzardo; vi è un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio che si occupa delle dipendenze, e sinceramente vorrei sapere cosa sta facendo - penso che prima o poi una risposta vada data in questa direzione - ed esistono le Regioni, cui è stato affidato il compito di cominciare a studiare i provvedimenti relativi

pensiamo anche alla vita concreta delle persone e ai servizi territoriali e *online* che possono curare, come succede nel mondo, tranne che in Italia perché qui è molto meglio ignorare il fenomeno o ricorrere ai grandi problemi invece di affrontare la quotidianità dei cittadini.

del gioco come intrattenimento nel gioco come possibilità di costruzione di una nuova vita. Noi non possiamo consentire che questa terribile illusione si faccia strada nei cittadini del nostro Paese. Occorrono campagne di prevenzione, di sensibilizzazione sull'uso del denaro e anche qualche scelta coraggiosa come, ad esempio, la carta del giocatore: una carta che sia come il codice fiscale del giocatore e che abbia un limite - ripeto, limite - di spesa, perché qualunque mercato ha un limite.

dipendenza che ha a che fare con la salute mentale. L'Organizzazione mondiale della sanità è stata chiara in materia: la salute, il benessere sono salute fisica e psichica. Non arriviamo all'ultimo momento, ad una serie di morti per usura, per gioco d'azzardo, per disperazione. Cerchiamo, una volta tanto, di porre in essere quella prevenzione che sola sola potrà contribuire in modo decisivo anche alla sconfitta di quel mercato illegale e terribile su cui speculano troppe persone nel nostro Paese. Per fare questo però occorre un patto

la legge *anti-gay* licenziata nei mesi scorsi dal Parlamento russo e firmata dal presidente Putin sancisce che la ''propaganda di relazioni sessuali non tradizionali davanti a minori'' è punibile con una multa che va dai 4.000 ai 5.000 rubli. Chi occupa una carica pubblica rischia una sanzione tra i 40.000 e i 50.000 rubli e uno straniero può subire anche l'espulsione o essere La legge estende a tutto il territorio nazionale una norma già in vigore a livello regionale a San Pietroburgo e in altre grandi città russe. D'ora in poi sarà reato parlare in pubblico dei diritti, degli amori e delle speranze dei cittadini gay. La definizione di propaganda darà al giudice la possibilità di punire con pesanti multe chiunque voglia parlare di diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali o transgender. si è creato nel mondo un vasto movimento di opinione pubblica che vuole sollevare questo tema, accompagnato anche da prese di posizione di Governi: penso ad esempio al ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle, che ha dichiarato che questa violazione dei diritti umani mette a rischio le relazioni tra Europa e Russia. Nella giornata del 3 settembre in diverse città italiane si sono svolte manifestazioni per chiedere una presa di posizione ai *leader* che si riuniranno nei prossimi giorni a San Pietroburgo. Il 5 e 6 settembre, Il 5 e 6 settembre, infatti, si terrà proprio a San Pietroburgo la riunione del G20, e tale consesso non può lasciare nel silenzio la grave violazione dei diritti umani in atto in questo momento in Russia. Il *premier* britannico David Cameron è intervenuto dicendo che in quei giorni solleverà la questione di fronte al Governo russo; il presidente Obama incontrerà a San Pietroburgo una delegazione di associazioni omosessuali. Ebbene, sarebbe molto utile - io ritengo che sarebbe necessario - che anche il Governo italiano facesse un gesto in questa direzione. Oggi il ministro degli esteri Emma Bonino è intervenuta criticando il criticando il gesto di Obama che a suo giudizio, in un momento di relazioni difficili con la Russia di fronte al caso siriano, rischia di irritare Putin; io ritengo però che non sia sia giusto, che non sia bene, che sbagli il ministro Bonino a mettere in contrapposizione la necessaria priorità di un'attenzione alla questione siriana con la necessità anche di rimarcare il rispetto dei diritti umani nello spazio europeo. Mi auguro quindi che il presidente del Consiglio Enrico Letta voglia cogliere questo appello ad unirsi a Cameron e a Obama nell'esprimere con un gesto, con un atto, anche la preoccupazione del Governo italiano per un balzo indietro di un grande Paese europeo come la Russia su questo tema; la Russia che solo vent'anni fa aveva depenalizzato il reato di omosessualità. un gesto che affermi la necessità del rispetto dei diritti umani come base necessaria delle relazioni internazionali fra i Paesi europei. *(Applausi

abbiamo tutti ricevuto un'*e-mail* da parte del Coordinamento comitati fuochi per evidenziare un fatto gravissimo avvenuto nei giorni scorsi. Mi riferisco alle dichiarazioni del camorrista collaboratore di giustizia Carmine Schiavone; ritengo però doveroso leggere questa nota qui in Aula: «Onorevole senatore, come lei ben sa, vaste aree della Regione Campania, in particolare i territori a nord di Napoli e a sud di Caserta, negli ultimi trent'anni hanno subito un'autentica, impietosa devastazione, soprattutto per il sistematico smaltimento illegale di rifiuti tossici provenienti dalle industrie del Nord e dal tessuto dell'economia illegale locale. Questa è una realtà incontrovertibile, accertata da Commissioni parlamentari e dagli organi giudiziari competenti, che solo chi è in malafede può negare. Intere popolazioni sono state così condannate, per i prossimi anni e per le future generazioni, a pagare, con la morte per cancro o con altre gravi patologie e malformazioni, lo smaltimento a "poco prezzo" di rifiuti tossici. Questo lucrosissimo "affare", tuttora in essere, è stato favorito anche da complicità e connivenze di esponenti delle istituzioni, alimentando la mancata gestione dei rifiuti urbani, perfettamente funzionale allo sviluppo del sistema criminoso. Proprio questa, nella nostra Regione, è stata addebitata a un popolo "brutto", "sporco" e "cattivo", irresponsabile ed ingovernabile, offrendo in questo modo un alibi perfetto per sommergerci di rifiuti industriali tossici. La cronaca degli ultimi giorni, con le dichiarazioni di uno dei protagonisti di questa realtà (il camorrista "collaboratore di giustizia" dal 1993 Carmine Schiavone), ha riacceso i riflettori sul terrificante e torbido scenario di crimini gravissimi, collusioni e complicità, che purtroppo tolgono credibilità alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Dagli stralci di interviste a Carmine Schiavone, trasmesse da Sky TG24 del 24 agosto 2013 emerge una realtà sulla quale è necessario che il Parlamento intervenga con assoluta urgenza. Carmine Schiavone afferma che, nelle Province di Napoli e Caserta, sono stati seppelliti fanghi termonucleari e tossici di vario tipo, anche con la complicità delle istituzioni dello Stato italiano preposte al governo e controllo dei territorio. Il Coordinamento comitati fuochi, che rappresenta circa 50 associazioni e comitati presenti sul territorio, chiede che vengano pubblicati tutti gli atti relativi alle dichiarazioni

Vi comunico, colleghi, di aver provveduto a richiedere all'archivio storico della Camera tutta la documentazione relativa alle audizioni effettuate nel 1997 dalla Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti che risultino ad oggi segretate. Spero vivamente che la suddetta documentazione possa essere disponibile agli italiani e comunico che noi del Movimento 5 Stelle, oltre a presentare un atto ispettivo, intraprenderemo ogni e qualsiasi azione per far luce e giustizia su quanto sopra esposto.

anticipato la collega Moronese, nei giorni scorsi l'ex collaboratore di giustizia Carmine Schiavone, uscito dal programma di protezione già da una decina di anni, ha rilasciato alcune interviste in cui ha reso delle dichiarazioni, in parte già note e discusse nei processi, in parte

tra le province di Napoli e Caserta, nelle zone del famoso comprensorio dei rifiuti, dove sono accatastate le ecoballe, e in tutte le campagne che furono della *Campania felix*, nonché in tutte le aree che sono state adibite a discariche di emergenza durante il periodo dell'emergenza rifiuti del 2007-2008, sono state rinvenuti centinaia e centinaia di fusti contenenti sostanze altamente tossiche

numerosi collaboratori di giustizia e in parte frutto di indagini autonome della magistratura e della polizia giudiziaria. Non sappiamo se esistano ancora dichiarazioni segretate di un certo valore rilasciate da alcuni collaboratori di giustizia. Mi consta personalmente, per aver partecipato a quelle operazioni, che numerosi interventi sono stati effettuati sul territorio, attraverso sistemi di ricerca molto sofisticati e anche molto costosi

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cito testualmente: «Una giornata particolare

Esultano per le neoplasie future degli abitanti di Parma, per il cibo avvelenato della Food Valley. Chi mangerà in futuro parmigiano e prosciutti imbottiti di diossina? L'inceneritore è inutile e brucerà rifiuti provenienti da ogni dove, ma loro sono contenti...».

Il fatto è che, per nostra sfortuna, chi dice queste parole dissennate è Beppe Grillo e la dichiarazione viene ripresa dai *media* di tutto il mondo. in tutto il mondo, si insinua il dubbio che il parmigiano-reggiano e il prosciutto di Parma siano imbottiti di diossina e che il "cibo avvelenato" della *food valley* generi neoplasie; demenziale e disastroso, un simile messaggio, per l'Italia, per Parma e provincia, parmigiani e parmensi, imprenditori e lavoratori del prestigioso sistema industriale alimentare. danno d'immagine e commerciale. Sulla dichiarazione stordisce il silenzio del sindaco di Parma, punta di diamante del Movimento 5 Stelle. La responsabilità della funzione avrebbe imposto ben altro atteggiamento: la difesa della sua città e la condanna, senza né se e né ma, delle parole del suo *leader* politico. Coraggiosamente, in altri casi, si è distinto e ha preso posizione; perché non in questo caso? Non può esserci questo silenzio e non c'è da parte dei parlamentari parmigiani. E non solo in nome dell'interesse della nostra zona, ma anche, in applicazione del principio dell'articolo 67 della Costituzione, nell'interesse della Nazione perché lo schiaffo e gli insulti al sistema produttivo alimentare italiano sono impliciti in questo messaggio, dato che Parma e la sua *food valley* ne fanno parte integrante e qualificante. Ringrazio la Ministro dell'agricoltura, onorevole Di Girolamo, per la tempestiva presa di posizione a nome del Governo. Mi auguro che, alla prima occasione utile, il presidente Enrico Letta voglia ritornare sul tema, magari con una visita nella stessa *food valley*.

sul fallimento della principale promessa elettorale del sindaco di Parma: quella di non di non far aprire il termovalorizzatore. *(Applausi

per fare in modo che questa riforma non cada sui propri passi, su alcuni aspetti sbagliati in essa contenuti e che abbiamo dimostrato in modo molto oggettivo e senza alcun campanilismo. Chiediamo che l'Aula discuta il disegno di legge già approvato in Commissione e si ponga fine ad una questione che rischia di diventare incresciosa e di creare imbarazzo nel rapporto tra il Parlamento e il Governo.

Il Governo, Presidente, come lei sa, ha uno strumento per correggere. Si tratta di un decreto correttivo previsto dalla stessa legge che aveva approvato questa riforma. Noi abbiamo avanzato una serie di proposte, tutte serie e condivisibili, pronte addirittura ad essere approvate all'unanimità. Ecco perché chiediamo

ricordo bene - e la Camera hanno approvato. Risulta alla Presidenza che ieri la Presidenza del Consiglio dei ministri si sia occupata della vicenda, avendo la possibilità di attuare

un efferato delitto è stato commesso questa mattina nella città di Bari. Vittima la dottoressa Paola Labriola, 53 anni, psichiatra, funzionario della sanità pubblica pugliese. Lascia il marito psicologo e due figli adolescenti. L'aggressione è avvenuta, come dicevo alle ore 9,30 nel quartiere Libertà di Bari: un quartiere difficile, signor Presidente. La dottoressa Labriola era testimone civile della difficile battaglia dello Stato sul fronte del *welfare*. Professionista integerrima della scommessa delle istituzioni nel campo del recupero e della cura delle patologie originate dal disagio sociale e causa, esse stesse, del disagio sociale nella dimensione individuale e collettiva. I colleghi di lavoro, i rappresentanti delle istituzioni cittadine e delle ASL, i familiari ed i pazienti, testimoniano all'unisono della grande abnegazione della dottoressa Labriola e del suo alto senso del dovere. Si parla, fra la gente del capoluogo pugliese, delle notevoli capacità professionali e umane della povera psichiatra assassinata. Una martire della psichiatra sul campo; una operatrice della sanità pubblica che dispiegava faticosamente i suoi effetti sul territorio. La dottoressa Labriola era sola nella sua opera professionale e nel mettere in gioco la sua vita? Godeva delle necessarie protezioni? Era al centro di un sufficiente sistema di sicurezza? Era bisognosa di attenzioni e di certezze nell'espletamento della sua preziosa azione quotidiana? Sono tutti interrogativi, signor Presidente, che ci sovvengono in mente per il ruolo e la funzione che esercitiamo in Parlamento a servizio del Paese e dei cittadini. Esprimiamo pertanto alla famiglia tutto lo sdegno per l'efferato atto e la solidarietà per la grave perdita. La dottoressa Labriola, fra l'altro, meditava il trasferimento dalla sua sede. Ella era in preda allo sconforto e, pertanto, tutti erano preoccupati.